L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Sull'ordine dei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 Comunico che, previ accordi tra i Gruppi e in relazione ad una concomitante cerimonia, la seduta di oggi si concluderà al termine della discussione generale del disegno di legge in materia di valutazione del comportamento degli studenti. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 23 aprile 2024, alle ore 12,30, con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Signora Presidente, onorevoli senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 924-*bis,* d'iniziativa del Governo, approvato dalla 7a Commissione permanente lo scorso 20 marzo. La Commissione, all'esito dell'esame in sede referente del testo risultante dallo stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, recante istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, è pervenuta alla definizione di un testo senza dubbio più ricco e completo rispetto a quello originariamente presentato, ma che, al pari del testo originario, si pone come obiettivo centrale quello di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti e riportando serenità nei rapporti tra studenti e insegnanti. Il disegno di legge proposto dalla Commissione risulta composto di tre articoli. All'articolo 1 permangono le disposizioni del disegno di legge originario in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Nello specifico, si interviene su un provvedimento normativo fondamentale in materia di valutazione del comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti, vale a dire il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge n. 107 del 13 luglio 2015. Tra le modificazioni apportate al suddetto decreto legislativo, segnalo quella relativa all'attribuzione del credito scolastico, ai sensi della quale il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzioni del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi. In materia di valutazione del comportamento, la Commissione propone l'inserimento di una disposizione di rilievo; il voto in condotta diventerà più influente e comportamenti violenti o aggressivi nei confronti di docenti, studenti e personale scolastico, che che determinano l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica, comporterà il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto. La mera sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, è infatti del tutto inefficace, anzi, può generare conseguenze negative sullo studente se non viene affiancata dalle suddette attività. La Commissione ha inoltre integrato i contenuti dell'articolo 1 con ulteriori disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti, prevedendo, con riferimento alla scuola primaria, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, mentre, per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, che la valutazione periodica e quella finale degli apprendimenti sia espressa con votazione in decimi. Nell'articolo 2

tenuto conto della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci. Infine, l'articolo 3, anch'esso formulato in sede di esame presso la Commissione, reca misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico. In particolare si prevede che con la sentenza di condanna per i reati commessi commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, sia sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. Signor Presidente, desidero iniziare questo intervento ringraziando innanzitutto il Governo e la sottosegretaria Frassinetti qui presente, che con impegno sta tracciando la strada per ridare alla scuola e ai docenti il ruolo che loro spetta, nell'interesse di uno sviluppo positivo, equilibrato e sereno dei ragazzi, affinché possano spendere proficuamente il periodo scolastico, per ottenere una formazione solida e competitiva. I giovani devono confrontarsi con una società complessa, dove non si può buttar via il tempo formativo a causa della irresponsabilità di minoranze influenzate ideologicamente. Desidero ringraziare anche il Ministro, che non perde occasione per valorizzare gli esempi positivi tra i ragazzi. Penso sia molto importante e dovremmo farlo tutti più spesso. E devo dire, colleghi dell'opposizione, che non l'ho mai sentito dalla vostra parte. Viviamo in una società dove l'aggressività è ovunque e dove i giovani non sfuggono al contagio; anzi, sono i primi ad essere investiti dai modelli negativi che imperversano. Pensiamo a fenomeni musicali quali quelli della *trap*, che inneggiano alla violenza, all'uso delle armi come *status symbol*, alla violenza nell'ambito della coppia e contro le donne, alle *fiction* e ai videogiochi, pieni di modelli negativi. Il rischio dell'emulazione è preoccupante. Quindi, deve essere forte e determinata la volontà di sostituire tali modelli con altri positivi. Il disegno di legge di cui discutiamo interviene con l'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, al fine di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, di affermare l'autorevolezza dei docenti, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire serenità all'ambiente di lavoro degli insegnanti del personale scolastico, per avere un percorso formativo degli studenti proficuo. Esso contiene delle norme molto significative, tra cui la responsabilità civile, azionabile direttamente dalla scuola nei confronti dei genitori che dovessero aggredire il personale scolastico. Di fronte ai ripetuti fenomeni di danneggiamenti nelle scuole e di aggressione nei riguardi dei professori e presidi, sia da parte degli alunni che dei familiari, di fronte alle sconcertanti immagini di scuole devastate, computer e lavagne sfasciati, immagini di teppismo e vandalismo allo stato puro, il Governo ha deciso di intervenire. Parliamo di situazioni che hanno inciso sulla serenità generale, che hanno privato migliaia di studenti del diritto allo studio per settimane a causa dell'azione di minoranze irresponsabili. Pertanto, il Governo ha deciso di porre in essere delle azioni chiare e concrete. Chi occupa e devasta una scuola merita il cinque in condotta e quindi la bocciatura. E la famiglia deve rispondere dei danni, perché non è giusto che la comunità si accolli anche i costi dei ripristini: è giusto che chi danneggia paghi. Allo stesso modo, il Governo ha voluto far sentire ai docenti la vicinanza dello Stato. Chi aggredisce un professore, infatti, aggredisce lo Stato. Quindi, non solo deve rispondere dei danni causati al docente, ma anche alla scuola, perché con l'aggressione viene messa in discussione l'autorevolezza della funzione educativa. è evidente che stiamo facendo i conti con le conseguenze degli errori del passato. Stiamo pagando gli eccessi ideologici del Sono necessarie, quindi, innanzitutto azioni concrete, come questa di cui discutiamo, chiare e dirette, per indicare ai giovani la strada. Ma serve anche una riflessione culturale. Bisogna ridare valore al principio di autorità. Quando un'autorità è legittima è un elemento essenziale per il funzionamento di uno Stato democratico; altrimenti, lo Stato finisce sotto la dittatura degli elementi eversivi, portatori di turbamento del vivere civile e onesto di famiglie e ragazzi, che con serietà si adoperano nella quotidianità. Quindi, occorre rimettere al centro il rispetto delle regole, così come bisogna affermare, proprio partendo dalla scuola, la cultura del rispetto verso la persona. Con questo provvedimento si va verso la giusta direzione; si dà peso alla funzione del voto in condotta e si rivede il sistema delle sospensioni, prevedendo una serie di attività, tra cui anche quelle di solidarietà sociale, proprio per stimolare il senso di responsabilità. Il ragazzo che sbaglia deve poter riflettere concretamente su cosa ha commesso, sul significato del senso di appartenenza alla comunità e sui doveri che ne discendono, perché crescere significa innanzitutto capire cosa sia la solidarietà e il rispetto del prossimo, per acquisire il concetto che non può esistere la felicità senza la responsabilità. Questo provvedimento rappresenta fattivamente il nostro desiderio di investire sui giovani, sulla costruzione delle generazioni future, dando loro le migliori condizioni per la crescita, innanzitutto scuole serene e funzionanti, affermando ogni giorno il ruolo centrale, educativo e sociale che la scuola deve ricoprire. Sarebbe significativo se tutta quest'Assemblea desse un segnale chiaro agli insegnanti, con un voto di sostegno e vicinanza, per dire che siamo con voi, siamo al vostro fianco e vicino ai ragazzi, per far vincere il bene. Noi di Fratelli d'Italia possiamo dire: siamo con voi, al vostro fianco, per dare alla scuola il ruolo che le spetta, per costruire una generazione vincente e positiva, condizione primaria per una Nazione sovrana e spiritualmente forte.

Signor Presidente, parto subito dalle ultime parole della collega Cosenza, che chiede a tutta l'Assemblea di esprimere grande solidarietà agli insegnanti, al loro lavoro e al fatto che tante volte sono vittime di un sistema che non li aiuta e che non gli è vicino. È successo Pioltello, per esempio: il sistema non è stato vicino agli insegnanti *(Applausi).* Mi auguro quindi

Il primo è il non fare differenza tra autorità e autorevolezza. La scuola e i nostri ragazzi i nostri ragazzi hanno bisogno di autorevolezza: ciò significa che hanno bisogno di figure adulte, capaci di dimostrare di essere adulte e di avere rispetto da parte degli studenti, perché gli studenti sono in grado di riconoscerli come figure capaci di essere di esempio e di manifestare pensieri forti che possano insegnare e aiutare loro a tirar fuori quello che sono. Diversa, dall'impostazione che è stata data da questo provvedimento, è l'idea invece di questo Governo: non è l'autorevolezza che deve emanare dalla figura dell'insegnante, ma è l'autorità, punto. È come se si partisse dal presupposto

Non penso che tutti siano buoni, ma penso che non esistano ragazzi cattivi; penso che esistano ragazzi con tutta una serie di difficoltà. Penso che, di fronte alle difficoltà educative, il compito di un educatore - perché l'insegnante è un educatore - sia quello di accompagnare,

si faccia così e non attraverso la paura. Non credo che l'idea del 6 in condotta possa modificare l'acquisizione di un percorso di crescita dei nostri ragazzi, che invece hanno bisogno di avvicinarsi a quel percorso accompagnati da persone nelle quali credono non per paura, ma per convinzione, perché ci credono, perché riconoscono in quelle figure gli educatori, cioè persone di cui fidarsi. Dire questo non significa essere lassisti o essere buonisti, ma significa dire che il rispetto delle regole lo si può avere attraverso la capacità di costruire una relazione basata sull'autorevolezza. Purtroppo non ci sembra che questo Governo abbia voluto costruire in questa direzione; sembra che basti un voto per cambiare la condotta e la condizione di una studentessa o di uno studente. Basta un voto: certo, che cosa c'è di più semplice del voto? Il fatto è che questo Governo crede veramente che basti un voto per cambiare le cose. Ci crede a tal punto che ha voluto eliminare, attraverso un emendamento, emendamento, una sperimentazione già in atto da tre anni con una valutazione descrittiva e formativa, sostituendola con qualcosa che, secondo il gergo e il linguaggio comune, "si capisce meglio". meglio". Infatti basta un voto per valutare la persona, no? Io, Presidente, non posso accettare questo tipo di pensiero. Non lo posso accettare perché credo profondamente nella professionalità degli insegnanti e perché, vede, nessuno di noi si sognerebbe di andare a toccare la carne viva del lavoro di un ingegnere, di un architetto, di un medico o di qualsiasi altro professionista.

in che modo devono valutare i ragazzi, perché così è più semplice e lo capiscono tutti. Vorrei fare allora degli esempi su come lo capiscono tutti. Presidente, mi rivolgo a lei. Immaginiamo di essere in una quarta della scuola primaria, quella che si chiamava scuola elementare, e di trovarci di fronte a una ragazzina o a un ragazzino che fa fatica a leggere, perché magari ha iniziato un po' più tardi, perché non tutti hanno gli stessi tempi. Questa ragazzina o questo ragazzino, attraverso un percorso fatto con l'insegnante, riesce a a raggiungere determinati obiettivi, che possono essere raccontati. L'insegnante gli può spiegare: «Guarda, sei partito da qui e siamo arrivati qui, devi essere contento, perché hai raggiunto dei grandi risultati». che chiaramente sono diversi da chi magari quella difficoltà nella lettura non ce l'aveva, perché partiva come un razzo (ripeto che i tempi sono diversi). Chiaramente l'insegnante valuterà, insieme a quella studentessa o a quello studente, il tipo di percorso e cercherà di dargli altri criteri. A questo servivano il voto descrittivo e la valutazione formativa: un voto che spiegava alle bambine e ai bambini, alle ragazzine e ai ragazzini da dove erano partiti, dove erano arrivati e su cosa avrebbero dovuto maggiormente concentrarsi insieme al loro insegnante, facendo un percorso insieme e soprattutto insegnando ai nostri bambini e alle nostre bambine che non sono un voto, non sono un giudizio, ma sono un percorso, perché sono in crescita. Questo era la *ratio* della valutazione formativa e descrittiva. È chiaro che può sembrare più difficile, perché la devi leggere, perché devi avere la pazienza di andare a vedere quello che l'insegnante ti sta dicendo, perché devi avere la pazienza, come genitore, di leggere tutti gli indicatori gli indicatori e di capire quali sono i progressi nella lettura, quali sono i progressi nella grammatica, in che modo puoi migliorare le tue competenze in un altro ambito, accompagnato, in una sorta di processo educativo quasi di reciprocità, perché la bambina o il bambino si sente accompagnato e l'insegnante che accompagna si trova investito della sfida di aiutare ogni singola alunna e ogni singolo alunno a raggiungere gli stessi risultati, pur partendo da situazioni diverse, valorizzando il percorso di ciascuno. La valutazione non è una cosa campata per aria; è una scienza, ci sono gli esperti, ci sono i pedagogisti, c'è chi lavora da tempo su ciò che è la valutazione. Non è semplicemente quel basta un numero, perché tanto io ti qualifico; c'è un percorso dietro, che questo Governo cancella e vuole cancellare con un emendamento, senza neppure porsi il tema che magari qualcuno avrà detto che questa è una valutazione difficile e che qualcuno si sarà anche lamentato.

per capire se questo tipo di valutazione ha portato risultati, visto che è in vigore da tre anni, in che modo le scuole hanno vissuto questo tipo di sperimentazione e cosa pensano gli insegnanti e anche gli studenti di questo accompagnamento. No: neppure nelle audizioni, perché questa idea e questo pensiero del tipo «tanto basta un numero, tanto basta un voto» a questa maggioranza sono venuti cammin facendo,

persone competenti che in tutto questo periodo, con pacatezza e modalità tranquilla, hanno provato a spiegare dove questa maggioranza stesse sbagliando. Quando è sorda, non danneggia solamente gli esperti della materia, ma soprattutto coloro che subiranno le ricadute di questa scelta, che è scellerata, perché farà male soprattutto

Ora, è chiaro che non possiamo attribuire il fatto che non vada tutto bene all'istituzione scolastica; abbiamo purtroppo fattori sociali complessi,

Un tempo i figli si facevano prima e c'erano comunità familiari composite: c'era la signora zia e c'era l'anziana nonna, che poteva aiutare nell'accudimento e ad indicare la strada; oggi invece, purtroppo, spesso la società porta i nostri bambini

tutti insieme per cercare di restituire all'istituzione scolastica quella grande capacità non solo di istruire, ma anche e fondamentalmente di educare. educare. Questa emergenza educativa è evidente a tutti, ne abbiamo parlato in seno alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e ne continuiamo a parlare. I professori, per esempio, e i maestri spesso hanno una concorrenza seducente e complicata da affrontare non solo per l'insegnante, ma anche per il genitore: vogliamo parlare dei *social media*, questi piccoli apparecchi che i nostri ragazzi possono tenere in mano ore ed ore, così pervasivi, influenti e forti nella capacità di incidere sulle loro coscienze? E da cosa sono guidati, da una volontà formativa ed educativa? Giammai, troppo spesso influenzati soltanto da logiche di tipo commerciale.

Prima qualcuno ha richiamato il tema del Ramadan. Esiste l'identità: nessuno vuole prevaricare l'identità altrui, ma sicuramente è importante che i nostri bambini siano cresciuti nella loro identità tradizionale. E allora il fatto di dire che ognuno possa celebrare il Ramadan come vuole non deve però implicare di vietare i bambini cristiani di poter frequentare la scuola. C'era un'insegnante importante, Maria Montessori, che diceva che per insegnare bisogna emozionare. emozionare. Il lavoro di questi insegnanti oggi è davvero molto complesso. Io, quando da genitore mi recai a prendere la pagella di mia figlia e lessi le valutazioni, rimasi un po' sbigottita. per esempio, lessi: «livello avanzato, l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note» (e già mi chiedevo quali fossero le situazioni note e quelle non note) «mobilitando una varietà di risorse fornite dal docente, reperite altrove».

Allora noi abbiamo queste quattro griglie, peraltro roteanti intorno alla mediocrità. Non c'è l'eccellenza e non c'è il cattivo voto. E allora io mi chiedo e vi chiedo: emozionano questo tipo di valutazioni? Emoziona forse di più prendere un 10 e lode? A me ha emozionato quando l'ho preso. Emoziona forse anche di più prendere un 2? Io credo di sì, perché io credo, senatrice Malpezzi, che non basti l'autorevolezza, ma serva anche l'autorità e se il bambino non ha studiato, se il bambino fa fatica, è bene che viva l'emozione di quel fallimento, perché questo lo aiuterà nella formazione del suo sé e della sua coscienza per migliorarsi. Io l'ho preso un 2, ho passato mesi per recuperarlo e lo ricordo. Mi è stato molto molto utile, mi creda. Oltretutto il genitore ha la capacità, visto che tutti noi siamo cresciuti con queste valutazioni, di comprendere meglio meglio l'*excursus* di questo ragazzo, quale sia la sua formazione. Quindi io sono vivamente convinta che questa sia la strada assolutamente migliore da percorrere. Oltretutto si tratta anche del tema della mancanza di rispetto della prima istituzione, spesso pubblica, con la quale i nostri bambini, che un domani saranno cittadini, entrano in contatto. contatto. È importante supportare adeguatamente gli insegnanti con tutti i provvedimenti che sono qui condensati. C'è una frase meravigliosa di papa Giovanni Paolo II, che disse che gli insegnanti italiani hanno alle loro spalle dei casi classici di esemplare attaccamento e dedizione alla scuola. Giosuè Carducci era professore universitario a Bologna; andò a Firenze per certe celebrazioni e una sera si congedò dal Ministro della pubblica istruzione. «Ma no», disse il Ministro, «resti anche domani». E lui rispose: «Eccellenza non posso, domani ho lezione all'università, i ragazzi mi aspettano». «Ma la dispenso io»,

C'è un'ultimissima postilla che vorrei aggiungere a questo discorso, e al riguardo voglio citare il Sottosegretario qui presente, che so avere grande sensibilità sul tema. Nelle istituzioni scolastiche oggi si è assistito a forme educative abbastanza discutibili. Stiamo vivendo la fase con il più basso tasso di natalità della nostra storia, e direi non solo italiana, ma anche europea. Credo che anche l'istituzione scolastica debba essere coinvolta in questo grande e complesso ragionamento, perché i bambini possono essere aiutati a comprendere il valore, un domani, oltre che di essere dei cittadini, di avere grandi responsabilità e di essere classe dirigente, magari dello Stato, anche di essere dei bravi genitori che accolgono la vita. quindi, che sarebbe veramente utile e valevole che si facesse un approfondimento, magari con il supporto di pedagogisti, di persone esperte, su come andare a supportare i nostri bambini, i nostri bambini, i nostri studenti degli istituti superiori, perché abbiamo delle stagioni molto complesse da affrontare e io credo che sia dall'educazione, dall'istituzione scolastica che si possono veramente creare i fondamenti della società dell'avvenire.

sulle modalità con cui valutare l'apprendimento degli studenti. Giustamente, ci sono sensibilità e proposte differenti e la valutazione si è fatta vieppiù precisa con riferimento sia alle conoscenze, sia alle competenze. Se è normale che vi siano, da questo punto di vista, sensibilità e proposte molteplici, credo che invece su un punto dobbiamo o almeno possiamo essere tutti d'accordo: la valutazione del comportamento. È chiaro che, accanto all'acquisizione di competenze e conoscenze, di qualità dell'apprendimento, la valutazione del comportamento, della responsabilità, della capacità di relazionarsi con gli altri, di vivere all'interno di una comunità in modo non conflittuale

dalle cronache dei giornali all'esperienza di ciascuno di noi, vediamo che i casi di aggressione nelle scuole sono aumentati e di molto - si parla di un aumento delle aggressioni superiore al 111 per cento - e i casi di insegnanti che vengono insultati e qualche volta persino attaccati dagli studenti sono davvero troppi. È evidente che nessuno si illude riguardo a questa situazione, nella quale si è frantumata una comunità educante, un'alleanza educativa tra la scuola che è fatta di insegnanti, personale, tecnico-amministrativo, studenti, e anche dalla famiglia. Di fronte famiglia. Di fronte a questa difficoltà, è chiaro che un atteggiamento sanzionatorio non sarebbe quello giusto. Eppure dobbiamo, da cittadini e genitori, essere consapevoli che un po' di terzietà

alla valutazione della condotta all'interno della valutazione complessiva degli studenti sia qualcosa che giova ai ragazzi, ma ovviamente a questa valutazione sia fatta non in maniera meramente sanzionatoria o punitiva, ma con un protagonismo degli studenti che hanno difficoltà nel comportamento. Mi spiego meglio. Con la collega Giusy Versace abbiamo presentato in Commissione degli emendamenti che sono stati approvati e che vanno nella direzione di rendere lo studente consapevole durante l'anno scolastico, laddove ci siano difficoltà nel comportamento, proprio per non arrivare alla bocciatura o alla sanzione, per consentirgli di prendere coscienza di comportamenti sbagliati e poter mettere in campo delle soluzioni. La collega Versace si è fortemente impegnata sul fronte di un ripristino di quel patto educativo il cui venir meno è la vera ragione dei fatti di cronaca cui tutti i giorni assistiamo, perché è chiaro che non si possono delegare alla sola scuola comportamento e l'educazione. Le famiglie devono avere una grande responsabilità e la delegittimazione del corpo insegnante, della funzione della scuola, è il primo errore che non dobbiamo fare da genitori e da cittadini, se vogliamo che che veramente quell'alleanza e quella collaborazione non si interrompano, ma possano funzionare. Ritengo pertanto che il provvedimento del Governo che reintroduce e ridà forza alla condotta vada nella direzione giusta. Così come penso si possa migliorare il sistema delle sospensioni. Oggi abbiamo il paradosso che il ragazzo che viene sospeso sostanzialmente viene ulteriormente allontanato dalla scuola. Invece, il fatto che all'interno di questo provvedimento si preveda che, laddove un ragazzo viene sospeso, si debba impegnare in un progetto di cittadinanza attiva, di inclusione sociale, di valorizzazione di un impegno che abbia una ricaduta utile per la comunità, è un modo per far sì che la sospensione non avvenga e non porti il ragazzo a stare a casa a guardare la televisione, ma sia un momento profondamente educativo. Ovviamente, se entriamo nel merito dei giudizi, capisco che ci possano essere sensibilità differenti, però dobbiamo trovare un'intesa almeno su un punto: quello di dare peso, di dare sostanza, di dare valore al comportamento e non solo all'apprendimento. La chiarezza sull'errore, su comportamenti eventualmente sbagliati, non è un modo per sanzionare o per punire lo studente: è un modo per metterlo nelle condizioni di condizioni di non diventare un bullo, di essere un domani un cittadino che ha rispetto della comunità, che si fa carico dei problemi della comunità. È anche un modo per costruire e ripristinare quell'alleanza tra la famiglia, la scuola, il corpo docente, che è alla base di una comunità educante che funzioni. L'ultimo punto è quello delle occupazioni. a questo, non possiamo far finta di non vedere quello che succede all'interno di tante e troppe scuole dove un conto sono i momenti di autogestione, che possono essere anche un momento di crescita, di confronto, nel quale si prova a trovare soluzioni, ci si interroga e si rendono gli studenti protagonisti nella soluzione di tante questioni organizzative o di studio. Un conto, però, sono le occupazioni che impediscono anche a chi non vuole occupare di poter andare a scuola e frequentare ed entrare nelle aule occupazionali che diventano una violazione di un servizio pubblico, oltre che un'interruzione di servizio pubblico. Io credo che questo sia un problema e far capire agli studenti il disvalore di tale comportamento è una nostra responsabilità.

dignità agli insegnanti e alla scuola non si può che essere tutti quanti d'accordo; dove, invece, c'è una divergenza profonda

si professa, come padre Zapata, la verità e poi si fa un cammino che è completamente diverso e che lo contraddice, perché è un testo che si fonda nella scelta strumentale privilegiata della repressione. Non c'è una parola dedicata alla prevenzione. La prevenzione si lega logicamente a un concetto di probabilità e vuole evitare che la probabilità si converta in una certezza negativa. La repressione, invece, agisce su una certezza negativa, storica, già avverata ed è la classica scorciatoia che si imbocca quando non si hanno la fantasia, la creatività, la volontà di innovare. La strada della prevenzione è una strada tutta in salita ed impervia.

La Corte costituzionale in numerose sentenze ci ha sempre spiegato che, anche se nella Carta non c'è un principio di ragionevolezza esplicitato, esso lo è nell'articolo 3 della Costituzione. Come diceva il grande costituzionalista Crisafulli, è un principio implicito, ma non pertanto meno efficace e meno stringente dei principi espliciti. Quindi, quando una legge professa un obiettivo e adotta degli strumenti che lo contraddicono, è una legge irragionevole che reca in sé un elemento di incostituzionalità. Questo va detto a chiare lettere. lettere. Noi non siamo assolutamente per le scorciatoie. Avremmo voluto almeno un minimo di attenzione alla prevenzione. Non c'è la previsione dell'investimento neanche di un euro bucato per quel che riguarda la formazione del corpo docenti. Come si può trasmettere agli studenti un'idea comportamentale corretta quando il corpo docente non è formato per questo? *(Applausi)*. È un'assurdità: si chiede al corpo docente un'impresa assolutamente impossibile. Tutte le riforme che sono state fatte di recente avversano questo risultato. È emblematico e significativo quello che è accaduto con l'ora di educazione civica. In questo modestissimo contenitore di un'ora settimanale ci abbiamo infilato tutto ed il contrario di tutto. È rimasta sempre un'ora

quando la folla si accalca per salire su un tram, faticosamente dal predellino riesce a entrare nell'abitacolo, intanto quelli che spingono da dietro finiscono per spingere quelli che sono davanti a loro, sicché escono dalla porta anteriore. Questo è quello che abbiamo fatto con l'ora di educazione civica. Ma dove vogliamo andare?

L'autorevolezza dell'insegnante è determinante nel conformare il comportamento dell'allievo, perché noi siamo per gli interventi conformativi e preventivi, non per quelli repressivi. Noi non siamo per la politica della clava:

Con la formazione, si affinano le metodologie e le strategie didattiche; mentre, senza formazione, l'autorevolezza diventa un sogno, una chimera, un traguardo difficilmente raggiungibile. Ripeto che questo Governo propone nella scuola - e non può fare diversamente - la rifrazione del suo modello di società: un modello autoritario, fondato sulla repressione, sulla politica della clava. Ciò si rifrange nel modello di scuola che viene proposto con questo disegno di legge. Ecco perché noi, che aborriamo i modelli autoritari, che siamo - secondo la celebre distinzione di Max Weber - per una democrazia rappresentativa, non plebiscitaria e autocratica, respingiamo questo modello di società e questo modello di scuola. e di dire che per noi è sempre un grande onore, un grande privilegio sedere con lei nei banchi di quest'Aula.

avete presentato questo provvedimento, sul voto in condotta e sul comportamento degli studenti, come al solito con un carico gigantesco di propaganda, sull'onda di episodi pesanti, anche drammatici, nelle nostre scuole. Lo avete fatto, però, in maniera assolutamente strumentale. Come a dire: adesso ci pensiamo noi, ristabiliamo ordine e disciplina come ai vecchi tempi; come a dire: buttiamo fuori dalla scuola un po' di studenti cattivi, e così tutto sarà risolto. Voi per primi, però, sapete che è solo scena. Questo provvedimento è inutile, perché sulla violenza a scuola bisogna intervenire a monte, per evitarla, e non a valle, per reprimerla, quando ormai è troppo tardi e le ferite rimangono e non cicatrizzano. Ed è un provvedimento dannoso, perché la valutazione che esaspera il peso del voto in condotta è una contraddizione in termini. È una valutazione che nega se stessa, perché sottintende un'idea repressiva e punitiva di scuola e quindi un'idea repressiva e punitiva di società. Siamo all'assurdo di un Governo che spaccia per riforma l'inasprimento del voto in condotta, cosa che, come tutti sanno, è completamente sbagliata dal punto di vista pedagogico. È il tentativo di un ritorno agli anni L'autorevolezza di un insegnante non si misura da un voto in condotta. *(Applausi).* Gli insegnanti sono i primi a saperlo: bocciature e sospensioni sono un fallimento, sono un *vulnus* per quella scuola dell'inclusione e dell'emancipazione che è scritta nella nostra Costituzione. voi rovesciate completamente la realtà. Puntate il dito contro gli studenti, alla fine come se fossero dei nemici, quando, invece, la missione della scuola è proprio mettere al centro i bisogni, le istanze e le aspettative degli studenti. Per voi tutto questo non esiste. Volete imporre un modello autoritario, per cui ogni contestazione potenzialmente è un reato. A voi non interessa che la scuola funzioni. A voi interessa trovare un capro espiatorio e criminalizzare una generazione. La date in pasto all'opinione pubblica come scansafatiche, degenerata, inutile, come la generazione *rave*, delle occupazioni, di quelli che sfasciano le scuole. In tal modo distogliete l'attenzione dal punto politico vero: noi abbiamo bisogno di sostenere le nuove generazioni, non di criminalizzarle, perché sono il nostro futuro. Abbiamo bisogno di fondi per il diritto allo studio, perché abbiamo dati insopportabili di abbandono e di dispersione scolastica che colpiscono ragazze e ragazzi delle famiglie più deboli e i territori più svantaggiati. La vostra è una politica, di fatto, di discriminazione sociale e, in alcuni casi, di feroce classismo. Povertà sociale e povertà educativa per voi non esistono e su questo non c'è nessun decreto. Eppure migliaia di ragazzi che vorrebbero continuare a studiare non possono farlo perché non hanno la possibilità economica, ma a voi evidentemente questo non interessa perché non porta consenso, perché non è facile da maneggiare come invece lo è un voto in condotta brandito sulla testa di chi organizza una manifestazione. Presidente, noi sappiamo bene quanto siano insopportabili il degrado o atti di violenza nelle scuole; lo sappiamo e sappiamo quanto sia difficile insegnare, stare in una scuola (faccio parte di una famiglia di insegnanti), ma la vertenza scuola non è una questione disciplinare, è una grande questione sociale. *(Applausi)*. Serve più scuola e servono più spazi; serve più tempo di apprendimento; servono più classi, con meno alunni; serve contrastare la precarietà asfissiante; serve contrastare il piano di dimensionamento che cancella intere scuole da luoghi dove ce n'è estremo bisogno; servono risorse per una scuola pubblica, aperta, inclusiva, progetti e passione che il Governo della destra invece mortifica. L'insegnamento si fonda su un patto di fiducia reciproca: lo sanno bene gli insegnanti. La responsabilità si fonda su un accordo reciproco. La comunità educante ha dimostrato durante il Covid di essere il perno della nostra società e sono sicuro che non accetterà questo tentativo di tornare indietro, perché minacce e autoritarismo cancellano decenni di conquiste e tradiscono un'idea sbagliata di società. La valutazione deve servire a rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e allo sviluppo: in questo senso riecheggia l'articolo 3 della nostra Costituzione. Voi invece fate l'opposto: con la valutazione create muri. Con i ragazzi bisogna discutere, avere la forza e il dovere di confrontarsi, perché esprimono una protesta che riguarda la scuola o il mondo in cui viviamo e vanno presi in considerazione. Voi invece stravolgete in questo atto lo statuto degli studenti, senza averli coinvolti. La scuola deve educare al pensiero critico, non reprimerlo. La critica e il conflitto sono il fondamento stesso della democrazia. Non è accettabile, come è successo a Modena, che un ragazzo, un rappresentante di istituto, che protesta e che pone una critica venga sospeso per dodici giorni: sono provvedimenti inquietanti. Pochi giorni fa, parlando di università, il presidente Mattarella le ha definite «luogo del libero dibattito, della critica e anche del dissenso nei confronti del potere». Presidente, penso che il sentimento di questa convinzione, espresso in maniera così nitida, riguardi in senso generale anche la nostra scuola, pur in contesti che sono molto differenti. Signora Sottosegretaria, c'è poi una norma in questo vostro provvedimento che contestiamo con forza ed è il ritorno al giudizio sintetico nella scuola primaria, quelle che erano le scuole elementari, la scuola delle bambine e dei bambini, l'età più importante e più indifesa, quella decisiva, secondo ogni pedagogista, per la crescita e la maturazione, per costruire fiducia in se stessi. Nel 2020, durante la pandemia, si è avviata una sperimentazione importante che ha coinvolto in questi anni scienziati, istituzioni scolastiche e famiglie. È stata introdotta una valutazione nuova, descrittiva, narrativa, cioè che racconta il bambino nella sua crescita, attenta ai bisogni dei bambini e delle diverse specificità; attenta al contesto sociale di partenza, che molto spesso è decisivo; attenta al fatto che ogni bambino è un mondo a sé, con tempi di sviluppo e apprendimento differenti che devono potersi esprimere senza barriere. Un bambino non può essere catalogato con un numero, con una lettera o con un titolo. La sua complessità deve essere colta e deve costituire il significato di una valutazione che non sia uno stigma, che non sia una macchia indelebile. Spesso un bambino o anche un ragazzo non è in grado di affrontare un brutto voto. E neanche la società lo è, fatemelo dire; una società che tende sempre più a discriminare. Il giudizio sintetico o, ancora peggio, il voto numerico hanno sempre una logica sommaria e sottendono sempre una logica punitiva. E ad essere puniti succede che siano sempre i bambini più svantaggiati e più fragili, quelli che vengono da famiglie in povertà. C'è stato un tempo, fino a non molti anni fa, in cui il voto che un bambino riceveva rimaneva quello per tutto il percorso scolastico, anzi per tutta la vita; un voto che per molti bambini è stata una condanna a non proseguire gli studi, quando invece sicuramente avevano tutte le potenzialità per farlo. Pensavamo di aver conquistato una scuola diversa, dove la valutazione non ha lo scopo di selezionare i migliori, ma di fare in modo che emerga, in tutti i bambini e i ragazzi, la loro parte migliore. Un giudizio di insufficienza per un bambino il più delle volte è fuorviante, blocca il processo di crescita formativa, non tiene conto dei livelli di partenza del bambino. La valutazione non deve classificare, ma raccontare un percorso personale, in cui c'è il mondo, ancora tutto da scrivere, di ogni bambino, un percorso cucito sulle reali possibilità di ogni alunno.

ma soprattutto per i bambini più deboli e per le famiglie più svantaggiate, perché il modello di valutazione presuppone un'idea di scuola, un'idea di società. Voi volete imporre un'idea sbagliata, autoritaria, gerarchica e punitiva, che separa anziché unire, che fa dell'errore uno stigma, mortificando bambini e ragazzi, privandoli delle loro motivazioni. Un provvedimento che aumenterà - ho concluso - dispersione e abbandono scolastico, impedendo a molti di continuare a studiare. Presidente, noi ci opporremo con forza e continueremo a batterci con

colleghi, signori del Governo, questo provvedimento ci convince moltissimo, in termini sia di merito, sia di di opportunità. Voglio ringraziare la relatrice, senatrice Bucalo, per il lavoro svolto. Credo si tratti di un lavoro assolutamente utile alla costruzione della società italiana del domani. credo che un provvedimento - come pure è stato detto da una parte delle opposizioni - che si pone come obiettivo centrale ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti, a non guardare le cose con una lente ideologica, che prescinda dalla realtà, sia qualcosa di assolutamente non criticabile. un provvedimento normativo che giudichiamo fondamentale, in materia di valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, che apporta una modifica importante al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con l'attribuzione del credito scolastico, ai sensi della quale il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportati nello scrutinio finale potrà essere attribuito solo se il comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi. In materia di valutazione del comportamento, la Commissione ha proposto l'inserimento di una disposizione di rilievo sulla base della quale l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporterà il coinvolgimento della studentessa o dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto. Si ritiene che la misura di sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, sia del tutto inefficace e, anzi, possa generare conseguenze negative sullo studente. Si prevede pertanto che la sospensione fino a due giorni dalle lezioni in classe comporti più scuola, più impegno e più studio. Lo studente sospeso sarà coinvolto in attività scolastiche assegnate dal consiglio di classe, di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. Qualora la sospensione superi i due giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterà le opportune coperture assicurative. Nel caso di sospensione superiore ai due giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo i principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Credo che quello che in realtà dice il testo sia profondamente diverso da quello che una parte dell'opposizione vuole far sembrare, perché nessuno vuole avallare la narrazione che la comunità studentesca sia di vandali e criminali. Chi lo dice questo? Chi lo ha detto? Nessuno lo sostiene. Quando però l'autorevolezza c'è e continua a mancare il rispetto, è importante affermare il ruolo dello Stato, perché il nostro corpo docente e tutto il personale della scuola rappresentano questa narrazione, che va assolutamente difesa, anche e soprattutto - a mio parere - nell'interesse degli studenti che sbagliano, ma possono rimediare. Nessuno crede che con un voto si possa risolvere la questione. Però credete in coscienza che la mancanza di tanti voti abbia determinato la situazione attuale? Mi sembra di ascoltare una costruzione e una narrazione tali per cui nella scuola italiana non ci sarebbe alcun problema e questo provvedimento finirebbe per rovinare tutto. A me non sembra una rappresentazione reale delle difficoltà che ci sono e che sono sotto gli occhi di tutti. Mi risulta poi abbastanza paradossale che una parte politica, che è stata ieri sostenitrice del 6 politico, oggi parli di autorevolezza e sia contraria al voto in condotta. Noi vogliamo governare il reale e sappiamo bene che nessuno è già promosso e nessuno è irrimediabilmente bocciato. Ma la guida è è lo Stato, quella cultura che vuole affermare che la libertà si costruisce attraverso il dovere.

fu rotto dalle fiamme, dalla distruzione e dalla morte, causata da un ignobile, vile attentato: litri di benzina fatti passare sotto la porta un innesco artigianale presso l'abitazione di una famiglia che aveva una sola colpa. Il padre, il rappresentante di quella famiglia, Mario Mattei, era il segretario della sezione del Movimento Sociale Italiano. In quegli anni prendersi la responsabilità di guidare una sede del Movimento Sociale Italiano in un quartiere popolare di Roma, come di tante altre zone d'Italia, significava essere minacciati tutti i giorni e rischiare quello che poi è successo quel giorno.

le altre figlie, Lucia, Silvia, la piccola Antonella, Giampaolo e gli stessi genitori, Mario Mattei e la moglie Annamaria, riuscirono

perché si sono sottratti alla giustizia, ma perché sono stati protetti e difesi da una controinchiesta (così si chiamava) che non rimase solo nel perimetro di quei gruppi della sinistra extraparlamentare, ma fu purtroppo purtroppo sostenuta e amplificata da molti esponenti, anche autorevoli, del mondo della sinistra e della cultura - spesso vengono citati da questo punto di vista Dario Fo e Franca Rame - essendo il clima di quegli anni di siffatto tipo.

Il modo migliore per rendere giustizia a Virgilio e a Stefano, ma a tutti coloro che sono caduti in quegli anni, di qualunque ideale, è che non parlino e che non parlino e non facciano più sentire la loro voce in quel modo i cattivi maestri di allora, che non hanno mai chiesto scusa alla famiglia per quello che hanno detto e per quello che hanno fatto e i cattivi maestri di oggi, che magari scrivono un libro, con poca empatia, per usare un eufemismo, verso altre vittime innocenti come quelli di Acca Larentia o che magari utilizzano la loro cattedra universitaria per inneggiare e per esaltare la lotta armata. *(Applausi)*. Ebbene, i cattivi maestri si facessero un esame di coscienza e rendessero onore alle vittime innocenti come Stefano e Virgilio Mattei. Grazie, Senato esprime dolore, voglio unirmi alle parole del senatore De Priamo, non foss'altro perché a me è toccato conoscere e abbracciare

Signor Presidente, come lei ha accennato, intervengo oggi in Aula perché vorrei anzitutto esprimere ufficialmente la nostra solidarietà per la recente aggressione al vescovo ortodosso avvenuta in una chiesa di Sydney nella giornata di domenica ed il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime della terribile aggressione avvenuta sabato scorso in un centro commerciale di Sydney. A loro esprimo la nostra vicinanza personale. Bondi Junction, signor Presidente, è un sobborgo a pochi chilometri dalla mia abitazione, una delle aree preferite dai nostri giovani emigrati, vicina alla famosa Bondi Beach, la spiaggia di Bondi, che lì hanno scelto di trasferirsi e spesso di avviare le proprie attività commerciali. Il centro commerciale Westfield è il punto d'incontro della locale comunità, giovani famiglie e anziani. Sabato era una tiepida giornata autunnale e migliaia di persone si trovavano nel centro commerciale, molti insieme ai loro bambini. Ho sentito in questi giorni amici che, signor Presidente, erano presenti o vicini al Westfield quel tragico pomeriggio di sabato e le assicuro che non si può che restare sconvolti nel sentire i loro racconti. Quanto accaduto è stato il folle gesto di una persona malata che ha ucciso sei persone e ne ha ferite oltre dieci, alcune ancora in condizioni critiche. Un gesto folle che ci ha ricordato quanto fragile possa essere la nostra quotidianità. Fra le vittime, una bambina di nove anni ancora in gravi condizioni in ospedale e la sua giovane mamma, che purtroppo non ce l'ha fatta. Cinque donne ed un uomo uccisi dalla follia di una persona sottoposta a cure psichiatriche. Si tratta di madri, figlie, studentesse ed un giovane immigrato che lavorava nel centro commerciale sottratti ai propri cari senza alcuna ragione o motivo. Questo tragico evento impone di riflettere su quanto anche noi qui in Italia facciamo per i problemi di salute mentale, se siamo efficienti nel riconoscere chi ha problemi e nell'accudirlo, se facciamo abbastanza per la sicurezza di chi vive quotidianamente questo problema e chi non sa di conviverci. La malattia mentale non è solo un problema individuale, ma sociale e va affrontato con attenzione e dedizione da parte delle istituzioni pubbliche, a partire dal Parlamento, che deve essere in prima linea nel riconoscerne l'importanza. Tramite lei, signor Presidente, mi appello al nostro Governo affinché mai si risparmi sulla sanità ed in particolare sui servizi di salute mentale. *(Applausi)*. Servizi che non solo aiutano gli individui a stare meglio, ma che sono fondamentali per prevenire conseguenze violente per se stessi e per gli altri. La seconda riflessione, avviandomi a concludere, signor Presidente, è relativa all'accesso alle armi da fuoco. Sono grato per la severità con cui la legge australiana regolamenta l'accesso a questi strumenti di morte;

Possiamo imparare tanto e se agiamo assieme per fare assieme un modesto passo in avanti per evitare che fatti del genere possano ripetersi, allora forse il sacrificio delle vittime di sabato scorso di Bondi Junction non sarà stato vano.

da qualche mese il Comune di Milano è salito alla ribalta delle cronache non per la solita immagine patinata della Milano da bere: pare che questa volta forse abbia un po' esagerato e l'immagine che la stampa e i *media* ci riportano non è esattamente quella di una città in piena forma. Infatti, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Beppe Sala è da mesi coinvolta in una serie di inchieste penali, insieme ai costruttori e gli operatori immobiliari, per i capi di imputazione di abuso edilizio, violazione di norme urbanistiche, lottizzazione abusiva,

La contestazione che viene avanzata è che invece, sulla base della vigente normativa, per edificazioni di questo genere, cioè per nuove edificazioni che non sono mere ristrutturazioni, occorre un permesso a costruire, con la correlata garanzia dell'erogazione degli standard e dei servizi ai cittadini (gli asili, il verde, le strade, i trasporti). inoltre che gli oneri di urbanizzazione siano stati monetizzati e quantificati in misura notevolmente inferiore al dovuto (circa un quarto del dovuto). Il problema non sono le norme, ma l'interpretazione che il Comune ne ha dato con determine e circolari interne. Il caso del Comune di Milano è un *unicum* in tutta Italia, cioè non c'è nessun altro Comune che abbia mai avuto un problema di questo genere, pertanto non c'è giurisprudenza né contrastante né univoca, quindi non è necessaria alcuna interpretazione autentica di queste norme. Non ci resta, quindi, che attendere l'esito dei giudizi. Nel frattempo il Comune si è mosso in autotutela, adeguando la lettura delle norme a quella comunemente utilizzata. Vorrei evidenziare in quest'Aula che in questa incresciosa vicenda mi pare che si stiano trascurando gli interessi dei cittadini, dei milanesi, che vedono sacrificati i propri diritti, sia dal punto di vista del danno erariale, sia dalla mancata erogazione dei servizi in misura adeguata. Infatti, se spunta un grattacielo di 80 metri con 300 famiglie, si devono anche garantire servizi commisurati per i nuovi insediamenti, ma questo non sta accadendo: dagli asili, che a Milano sono drammaticamente insufficienti, al verde, bene raro, prezioso e insufficiente. A Milano abbiamo, infatti, la più bassa quota di verde *pro capite*, sotto il livello della media e questa vicenda accade proprio in una città che ne avrebbe bisogno come l'aria, come l'aria pessima che siamo costretti a respirare: a Milano ogni anno muoiono 3.000 persone a causa dell'inquinamento dell'aria. Questo verde, che manca e che non è previsto in questi interventi, andrebbe a migliorare la qualità dell'aria, come anche a mitigare il fenomeno delle isole di calore che arroventano giorni e notti a Milano. Insomma, il mio auspicio è che ci si preoccupi più di una Milano da vivere

Signora Presidente, questa è la storia di una donna a cui hanno diagnosticato due anni fa il cancro al pancreas. Attraverso la sua storia capiremo l'importanza delle Pancreas *unit*. Mi scrive Clotilde: ho un piccolo cappellino di stoffa al posto dei miei biondi capelli. Curavo le mie chiome tutte le sere, lo facevo perché al mattino mi piaceva vedere queste onde di capelli incorniciare il mio viso diafano e sorridevo, per un attimo, con i miei occhi verdi, di un verde profondo come quello dei mari esotici di una cartolina, oggi diremmo di un *reel*. All'inizio ero molto spaventata dalla diagnosi. Tutti sanno che il cancro al pancreas è molto complesso da affrontare e ha un'alta mortalità nonostante le cure, anche perché spesso è diagnosticato molto tardi. Ho trovato dei centri però in Italia che affrontano le cure, ma purtroppo non dovunque nello stesso modo, con la stessa possibilità di sopravvivenza. Non avevo scelta però e sono andata al Nord dove avevo compreso che ci sarebbero state migliori possibilità di cure. Ho fatto tutto, ho accettato il mio destino. Ci vuole un coraggio enorme ad affrontare questa malattia, ma anche la morte a eppure non mi sono mai vista vecchia, ma non auguro a nessuno di vivere in questo modo. Ho provato anche una terapia sperimentale, che offre 1,9 mesi di vita in più. Quando sai che l'aspettativa di vita è breve, un mese ti sembra un anno. La terapia però, almeno su di me, non ha funzionato e le mie condizioni si sono aggravate. Adesso sono qui in una terapia intensiva di un ospedale pubblico della Campania e ho deciso di tornare qui perché, per un miracolo, per una coincidenza, qui lavora mia sorella anestesista. Io non so quanti altri giorni o mesi mi restano da vivere, ma voglio affrontare la vita che mi resta con tutto il coraggio con cui ho affrontato la vita di tutti i giorni. Ho voluto raccontarvi la mia storia per darvi coraggio, per infondere a tutti voi il coraggio di trovare una soluzione alle Pancreas *unit*. Io so bene che è difficile fare questo, ma ho chiesto ad Orfeo, al senatore Mazzella, al mio caro Orfeo, di interessarsi insieme con il senatore Zaffini affinché si possano realizzare queste Pancreas *unit* in modo da distribuire in modo uniforme in tutta Italia delle unità operative. Dovete sapere che le opzioni terapeutiche attualmente disponibili per questo tipo di cancro sono la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia, ma - ripeto - non sono disponibili con la stessa qualità di cure in ogni Regione e nel 2023 sono state stimate circa 14.800 nuove diagnosi. Si tratta di uno dei pochi tumori che risulta in aumento per incidenza di mortalità in tutte le fasce di età. età. Permettetemi perciò di ringraziare ancora la 10a Commissione, il presidente Zaffini, ma anche l'associazione Codice viola e Piero Rivizzigno, care senatrici, cari senatori, la possibilità di dare a noi, malati di cancro al pancreas, qualche mese di più, qualche anno e, magari un giorno, le cure definitive. Grazie senatore, per aver condiviso con noi questa storia. Esprimo la nostra vicinanza a tutti i malati oncologici che in questo momento stanno combattendo questa battaglia.